Care senatrici, cari senatori, sapete già che ieri si è spenta, all'età di ottantanove anni, la signora Clio Maria Bittoni, moglie dell'indimenticato presidente emerito Giorgio Napolitano. Io ho avuto l'onore e il piacere di conoscerla e di incontrarla spesso durante gli anni in cui ho ricoperto immeritatamente l'incarico di Ministro della difesa. Ho potuto di persona rilevare come fosse una donna risoluta e rigorosa, ma anche sobria e sempre ironica, esattamente come la descrivono stamani tutte le persone che la conoscevano bene. Il suo ricordo mi è rimasto molto impresso nella memoria per la capacità che aveva di essere sempre presente con il marito senza mai apparire, sempre alle spalle, ma sempre importante per lui. Io ho avuto questa netta impressione che mi viene confermata da coloro che le sono stati più vicini.

ci uniamo nel triste ricordo. Molti oggi raccontano aneddoti della sua vita; quella volta che venne investita da un'auto, mentre da sola, come una normale cittadina, attraversava la strada davanti al Palazzo presidenziale, e poi, quando si mise in fila per acquistare personalmente il biglietto di una mostra allestita nelle Scuderie del Quirinale, lei, moglie del Presidente. forse questi due aneddoti ne danno la dimensione e la misura più di tante altre parole. Una donna, quindi, che possiamo definire semplice e amabile. Questo e tanto altro ancora è stata la signora Clio Napolitano, che ora torna di nuovo a fianco di suo marito Giorgio, così come lo è stata ininterrottamente dal 1958, anno in cui si sono conosciuti, fino alla scomparsa del Presidente avvenuta, come sapete, il 22 settembre 2023. Invito il Senato a osservare qualche istante di raccoglimento in ricordo della signora Clio Maria Bittoni.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

ci tengo in modo particolare a prendere la parola oggi non solo per ringraziare, ma per complimentarmi e chiedervi di unirvi ai miei complimenti per tutti gli straordinari successi ottenuti a Parigi dai nostri atleti olimpici e paralimpici. Trovo doveroso farlo in quest'Aula, Presidente,

anche al presidente Marti che si è fatto portavoce e ha suggerito questa missione; mi avete dato l'onore di potervi rappresentare per raccontare quanto l'Istituzione sia vicina al mondo paralimpico. Ed è stata anche l'occasione

che merita invece di essere sostenuto. Un grande plauso va non solo a tutti gli atleti, ma anche a tutti i tecnici, alle federazioni, ai gruppi sportivi, all'impegno che ci mettono i presidenti Malagò e Pancalli, ma anche al contributo che dà l'azienda sport e salute. È un gioco di squadra: quando trionfiamo e sventoliamo il Tricolore, lo facciamo anche grazie al fatto che alla base c'è un grande lavoro di squadra. Qualcuno più importante di me disse in tempi non sospetti che lo sport

Tutto questo ha permesso anche di raccontare le nostre storie, che possono essere di stimolo anche per altri, per coloro che ci guardano. Sono felice felice del fatto che quest'anno l'attenzione così elevata abbia contribuito anche ad ottenere un cambio culturale necessario, un approccio approccio decisamente diverso e migliore nei confronti di chi vive con una disabilità. Spero che questo tipo di integrazione che si respira all'interno di un campo d'atletica e all'interno del mondo paralimpico si possa respirare dappertutto, nelle città, nelle metropolitane, nei Comuni, nelle scuole, nei luoghi di lavoro. La ringrazio, signor Presidente, per avermi dato questa opportunità. Spero di avervi rappresentato al meglio,

Posso confermare che siamo veramente orgogliosi di essere stati rappresentati da lei alle Paralimpiadi. Siamo davvero tutti orgogliosi.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 3 ottobre. La seduta di oggi prevede la discussione di ratifiche di accordi internazionali e le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, sui disegni di legge collegati su semplificazione e digitalizzazione di attività economiche e servizi e in materia di semplificazione normativa e qualità della normazione. avranno luogo il sindacato ispettivo la mattina e, alle ore 15, il *question time* con la presenza dei Ministri degli affari esteri, delle infrastrutture e dell'istruzione. Il calendario della prossima settimana prevede la discussione del disegno di legge, dalla sede redigente, sulla morte medicalmente assistita redigente, sulla morte medicalmente assistita e del disegno di legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Per quest'ultimo provvedimento gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 10 di domani. Nella settimana saranno inoltre discussi, dalla sede redigente, i seguenti disegni di legge: norme in tema di legittimo impedimento del difensore; istituzione della Giornata nazionale del formatore; agevolazioni fiscali *start-up*; organizzazione del Macerata Opera Festival. 18 settembre, alle ore 15, verrà discussa l'interpellanza a procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, sull'impatto derivante sui conti pubblici dall'attuazione dell'autonomia differenziata. Nella settimana dal 24 al 26 settembre lavori prevede, oltre a eventuali argomenti non conclusi, la discussione del decreto-legge in materia di misure di carattere fiscale ed economico. Giovedì 26 avrà luogo la votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di amministrazione della RAI. La settimana dall'1 al 3 ottobre sarà riservata alla discussione di eventuali argomenti non conclusi. Giovedì 19 e 26 settembre e giovedì 3 ottobre avranno luogo il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*. Il calendario sarà integrato

è convocato martedì 17 settembre, alle ore 12,30, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

comunicazioni al Senato martedì 15 ottobre, alle ore 15, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021, di seguito denominata « Convenzione ».

l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Repubblica del Kosovo per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali. Sottoscritta dall'Italia e dal Kosovo nel giugno 2021, la Convenzione oggi al nostro esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, prevenire le evasioni fiscali e porre gli investitori italiani in una posizione concorrenziale rispetto agli operatori economici di altre nazionalità. L'intesa richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti, limitandone all'imposizione sui redditi e, per la parte italiana, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società e all'imposta regionale sulle attività produttive. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Signor Presidente, annuncio che interverrò soltanto in questo caso e rinunciando ai due interventi successivi perché le considerazioni sono le stesse. Voteremo favorevolmente. Si tratta di accordi che, ovviamente, la Repubblica italiana conclude con quanti più Stati possibili, perché vanno a semplificare il rapporto tra il cittadino e il fisco. Sono anche rivolti alla riduzione dell'elusione e dell'evasione fiscale. Quindi, non c'è nessuna ragione per non votare a favore. Si tratta anche di accordi fatti da Governi di vario colore e di vario orientamento, a dimostrazione che si tratta di un orientamento condiviso. Anche le votazioni che abbiamo visto finora, per cui l'intero Senato ha votato favorevolmente, vanno in quella direzione. Quindi, sia per questo disegno di legge di ratifica che per i due successivi che affronteremo quest'oggi, il voto del Gruppo Italia Viva sarà favorevole.

dei Paesi che firmano la convenzione, per garantire gli investimenti diretti e soprattutto le attività imprenditoriali negli altri Paesi, in un clima di maggiore di maggiore chiarezza. In questo caso, nei confronti dello Stato libico un vecchio accordo, fatto già nel 2009, ai tempi del Governo Berlusconi, che poi non aveva potuto vedere il procedimento di ratifica, per la mancanza di atti da parte del Governo libico, perché arrivarono le cosiddette primavere arabe,

diventato poi Stato libico, e oggi siamo pronti, insieme alle altre convenzioni con il Kosovo e con la Repubblica popolare cinese, a ratificare una serie di accordi che mancavano per dare un quadro normativo più chiaro negli scambi internazionali, nelle attività imprenditoriali e sugli investimenti diretti. Da questo punto di vista, lo schema è lo stesso di quello con la Repubblica del Kosovo. Con riferimento agli oneri economici, dall'attuazione dello strumento di ratifica

Signor Presidente, oggi ci troviamo a votare la ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato della Libia in materia fiscale. Questo accordo rappresenta un passo significativo nella nostra cooperazione internazionale e nel rafforzamento delle relazioni economiche tra i due Stati. La Convenzione non solo si applica ai residenti di entrambi i Paesi, ma affronta anche questioni fondamentali legate alle imposte dirette e alla non discriminazione fiscale. cruciale che i cittadini e le imprese italiane e libiche possano operare in un contesto di certezza e trasparenza e questa convenzione offre garanzie in tal senso. Uno dei punti più salienti è la definizione di stabile organizzazione, che ci consente di stabilire in modo chiaro le condizioni in cui uno Stato può esercitare la propria potestà impositiva e questo - è importante sottolinearlo, come ha fatto il relatore Alfieri - è in linea con gli *standard* dell'OCSE. In questo accordo manca qualcosa che avremmo voluto e io ho fatto un intervento in questo senso anche nella 4a Commissione

situazioni sicuramente importanti e di vantaggio, in alcuni territori come quello libico che sappiamo non essere pienamente controllato dallo Stato, possano rischiare di andare a vantaggio di organizzazioni che purtroppo ledono in maniera massiva i diritti umani e i diritti fondamentali. Pertanto introdurre una clausola di condizionalità, come del resto si fa di sovente nell'Unione europea, credo possa essere una garanzia perché gli italiani sappiano che questi vantaggi vanno ai cittadini e alle imprese, e che nessuna delle risorse pubbliche dello Stato italiano può essere direttamente o indirettamente collegata a episodi di violazione dei diritti umani. nostra sottolineatura, noi riteniamo che, per i motivi legati alla cooperazione amministrativa e alla cooperazione fiscale, sia importante approvare la Convenzione. Per questo il Gruppo Azione voterà favorevolmente.

oggi votiamo la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire l'evasione fiscale. Il testo, basato in larga parte sul modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, si applica ai residenti di entrambi gli Stati e riguarda le imposte dirette elencate e, per quanto riguarda il principio di non discriminazione e gli aspetti di cooperazione amministrativa, le imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche e/o giuridiche. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dalla nostra Nazione. Annuncio così il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

nella *Gazzetta Ufficiale*. DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. L'Accordo in via di ratifica intende porsi quale aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta e nelle relazioni economiche e fiscali tra le due Nazioni, adeguandone le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali e in particolare assumendo a modello la Convenzione elaborata nell'ambito dell'OCSE. Esso è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale. L'intesa bilaterale, una volta entrata in vigore, consentirà così alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende delle altre Nazioni europee, nonché agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in circa 10,86 milioni di euro a decorrere dal 2025. È per questi motivi, in conclusione, che si propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

molto chiare e, a mio parere, soddisfacenti alla Camera dei deputati. Assistiamo all'ennesimo colpo di mano di Maduro. Assistiamo all'umiliazione di qualsiasi speranza democratica. Assistiamo alla persecuzione di un'opposizione che si incarna in persone

È stato prelevato e la sua famiglia, a distanza di un mese e mezzo, non ha ancora avuto la possibilità di incontrarlo. Sembra che sia in un carcere di massima sicurezza, laddove vengono perpetrate le peggiori iniziative da parte del regime. Io ritengo importante che il Parlamento italiano, il Governo italiano e le forze politiche tutte intervengano, perché qua non c'è destra o sinistra che regga, ma c'è l'Italia, con la sua credibilità democratica, che deve richiedere l'immediata scarcerazione di un suo concittadino, Américo de Grazia, e di quanti sono come lui perseguitati. È un momento terribile per quel Paese. Noi, con la presidente Craxi, abbiamo seguito la vicenda in Commissione esteri e abbiamo anche dato credito al processo elettorale, sperando di poter arrivare a una qualche soluzione, dopo anni di angosce per quel popolo, un popolo che non le merita, un popolo che agli inizi degli anni Settanta era tra i popoli più avanzati del pianeta. Si andava a investire in Venezuela, perché il risultato era praticamente assicurato. oggi quel popolo subisce un'umiliazione e un oltraggio quotidiano. Nell'esprimere solidarietà ai democratici venezuelani, rinnovo l'invito perché il Governo e il Parlamento si muovano immediatamente, tramite le nostre rappresentanze diplomatiche, per chiedere che sia che sia assicurata la libertà per Américo de Grazia e per i prigionieri politici. ringrazio il senatore Casini. Come egli giustamente ha detto, io da questa parte dell'Emiciclo e lui dall'altra seguiamo con attenzione il dramma del popolo venezuelano. La Commissione esteri del Senato si è già mossa in questo senso. Ieri ho personalmente investito l'ambasciatore De Vito sul caso de Grazia;

Signor Presidente, è stato un agosto torrido non solo per il clima metereologico, ma anche per il sistema delle relazioni fra di noi componenti di questa Assemblea e sul piano delle relazioni politiche. Nel quadro di questa situazione vorrei sottolineare due aspetti per quanto riguarda il primo aspetto, voglio dare atto alla Presidenza tenuto conto del fatto che questo agosto torrido ci ha costretti a rivolgerci inusualmente per tre volte, attraverso delle missive, al Presidente del Senato

la Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente del Senato, abbia deciso di richiedere, attraverso lo strumento del *question time*, la presenza della *premier* Meloni all'interno di quest'Aula, con riferimento alle vicende di questo agosto,

i rapporti fra di noi e anche le modalità con le quali esprimiamo le nostre relazioni. Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'inizio di agosto, la nostra collega Raffaella Paita, coordinatrice del nostro partito, e un'altra collega della Camera, l'onorevole Maria Elena Boschi, hanno svolto una funzione di sindacato ispettivo che rientra in pieno all'interno delle prerogative assegnate a ciascun parlamentare. Non hanno fatto attacchi personali, non hanno introdotto elementi spuri all'interno del dibattito: hanno fornito una serie di elementi specifici, che rientrano in pieno nell'ambito delle loro competenze, delle loro prerogative e - aggiungerei - anche dei doveri dei parlamentari, quantomeno dei parlamentari delle opposizioni. Per aver svolto questa funzione, hanno ricevuto, prima la senatrice Paita e, poi, le colleghe del Gruppo che io ho l'onore di presiedere, una serie di epiteti da parte di alcune componenti di questa Assemblea. Signor Presidente, chiedo a lei se sia normale definire dei colleghi che fanno il loro lavoro una muta di cani. È normale, secondo lei, definire un membro della nostra Assemblea, che ha svolto anche l'alta funzione di Presidente del Consiglio, un boss fallito di Provincia, un capobranco o ancora un padre padrone?

degli «strumenti arrendevoli del maschio padrone che si nasconde alle loro spalle»? Secondo noi, no. Noi vogliamo fare un appello affinché si riconduca il nostro dibattito non solo a una normale educazione, ma anche a una maggiore continenza verbale e al rispetto di tutti i colleghi parlamentari. Se si ha la concezione che la politica è tutto, allora ci si sente in diritto di fare e di dire tutto. Se invece si ha la coscienza che la politica, esattamente come altri esercizi umani, ha un limite, allora a quel punto esiste un limite che non può e non deve essere superato. Noi crediamo che nella circostanza questo limite sia stato superato e, nel manifestare la mia solidarietà alla senatrice Paita e a tutte le senatrici del mio Gruppo, chiedo che la Presidenza in futuro si possa fare garante che questi elementi vengano assicurati anche nel prosieguo della nostra attività parlamentare.

«Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese». Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente,

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che le risoluzioni approvate dai due rami del Parlamento nelle sedute dell'11 ottobre 2023 sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 hanno aggiunto, tra i disegni di legge da considerare collegati, il seguente provvedimento «Disegno di legge per la semplificazione e la digitalizzazione dei provvedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese». Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 5 luglio scorso. Per quanto riguarda i requisiti della rispondenza agli obiettivi programmatici e della omogeneità, di cui all'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009, si osserva che il disegno di legge in esame risulta composto di 33 articoli, distinti in quattro Titoli: il Titolo I recante "Misure di semplificazione delle attività economiche", a sua volta distinto in quattro Capi, relativi rispettivamente alle imprese, al turismo, alla navigazione e a ulteriori misure di semplificazione; il Titolo II recante "Misure di semplificazione in favore dei cittadini", distinto in due Capi, relativi rispettivamente ai procedimenti amministrativi in favore dei cittadini e alla materia dell'istruzione; il Titolo III recante "Ulteriori misure di semplificazione", distinto in quattro Capi, relativi rispettivamente all'università, alla materia sanitaria, alla pubblica sicurezza e all'attuazione degli obblighi di legge; infine, il Titolo IV recante "Disposizioni finali". In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nelle suddette risoluzioni di approvazione della NADEF 2023, ad eccezione dell'articolo 23, recante: "Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025", che risulta estraneo all'oggetto.

e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 1184 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente, e risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione dell'articolo 23. Dispongo pertanto lo stralcio della predetta disposizione, che andrà a costituire l'autonomo disegno di legge n. 1184-*bis*, recante «Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025». L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1192 recante: «Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie». Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2024, come approvato nella risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha tra l'altro confermato quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico, ossia nella NADEF 2023. Quest'ultimo Documento ha indicato, tra i disegni di legge da considerare collegati, anche il seguente provvedimento: "Misure in materia di semplificazione normativa". Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 15 luglio scorso. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023. Il provvedimento, composto di 12 articoli, distinti in quattro Capi, appare inoltre coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni risultano quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica». Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 1192 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente.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

esattamente a quest'ora, il 9 settembre 1944, alla periferia di Domodossola si completava la trattativa fra i capi partigiani delle Brigate Valdossola e Valtoce e l'esercito di occupazione nazista e la milizia fascista per la liberazione delle Valli dell'Ossola e della Valle Cannobina. Nasceva così quella che verrà ricordata come la Repubblica libera e partigiana dell'Ossola, oppure, dal punto di vista più comunicativo, i quaranta giorni di libertà. Fu un'esperienza nella quale, nel cuore della drammatica esperienza bellica della Seconda guerra mondiale, nel nostro Paese forze militari e popolo si univano per giungere a una liberazione e all'affermazione che la libertà e la democrazia dovevano tornare a essere l'elemento fondante per la ricostruzione della trama nazionale. Credo sia giusto e doveroso, signor Presidente, sottolineare questi elementi e codesta ricorrenza, soprattutto in connessione con il ruolo che la Repubblica dell'Ossola ebbe nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente. Come ebbero modo di ricordare, fra gli altri, Sandro Pertini e Aldo Moro, l'esperienza della Giunta dell'Ossola (composta esclusivamente da persone non militari perché i militari, una volta raggiunto il potere,

tre componenti di questa Assemblea furono tra i protagonisti di quell'esperienza. Penso al presidente della Giunta provvisoria di Governo, professor Ettore Tibaldi, peraltro originario proprio del pavese, da cui lei proviene, signor Presidente, sfollato nella Valle dell'Ossola e che ebbe il coraggio, insieme con il segretario generale di quell'esperienza, che presiedette l'Assemblea costituente, Umberto Terracini, di tradurre in atti amministrativi quelle esperienze. Ricordo anche due senatori: il senatore Francesco Albertini del Partito Socialista, che per essere tra gli organizzatori della Repubblica dell'Ossola finirà a Mauthausen, e la medaglia d'argento Fausto Del Ponte, che poi verrà su questi banchi per due legislature. Sono tutte persone che possono costituire oggi, insieme con le donne e gli uomini che parteciparono a quella straordinaria pagina, un esempio, un modello e un richiamo ai valori che

che preoccupa e che - credo - debba preoccupare fortemente coloro che si occupano più direttamente di diritti umani in Europa, nei Paesi non parte dell'Unione europea, ma sicuramente Paesi europei come la Bielorussia; si preoccupano della repressione contro i prigionieri politici da parte del regime di Lukaschenka in tutti i modi e del processo di debielorussizzazione della cultura di quel Paese, di quel popolo, che continua in un modo atroce e che deve essere conosciuto dall'opinione pubblica politica e ottenere l'appoggio a livello parlamentare, nei confronti dell'opposizione, del Gabinetto unitario di transizione. È giunta notizia che una grande musicista, *leader* del movimento di opposizione, sostenitrice della presidente Svjatlana Tsikhanouskaya - la chiamo Presidente perché è colei che quattro anni fa aveva realmente vinto le elezioni, poi rubate da Lukaschenka - *Maria*

nella prigione nella quale è detenuta da quattro anni. Non è evidentemente la sola a subire una tale sorte, perché sono più di 1.500 i prigionieri politici nelle carceri del regime bielorusso.

numerose decine di più ogni volta che si fanno queste operazioni di presentazione per l'opinione pubblica. La collaborazione e la cooperazione con il Governo unitario di transizione è un fatto acquisito da parte del Parlamento europeo che, non più di un anno fa, ha scritto una lettera di intenti formale per collaborare nello scambio di informazioni, nell'azione che possa sostenere l'opposizione in Bielorussia. Nella stessa direzione si sono posti gli Stati Uniti e si stanno ponendo il Canada e la Nuova Zelanda. lancio un appello in questa sede e un invito, affinché i colleghi che si interessano più direttamente di tali problematiche all'interno di questa Camera e del Parlamento si impegnino nel gruppo "Amici

Signor Presidente, ringrazio e mi associo alle parole del presidente Terzi sulle condizioni di detenzione in Bielorussia, nella colonia penale di Gomel, di Maria Kalesnikava, una delle *leader*, accanto alla citata Svjatlana Tsikhanouskaya, della resistenza democratica contro l'atro regime di Lukaschenka, il servo di Putin. Secondo testimonianze dirette di detenuti, la Kalesnikava sarebbe arrivata a pesare poco più di 40 chili: una donna alta un metro e settantacinque, asfissiata in un regime di isolamento totale dal resto del mondo, in una pena che somiglia a un assassinio per fame. La sorella, T*atiana* Khomich, ha denunciato questo gravissimo ed insopportabile sopruso, la mancanza di notizie sulle sorti di Kalesnikava, e lanciato una campagna di sensibilizzazione internazionale, SOS Maria, perché da più parti venga la richiesta di notizie e rassicurazioni di fronte a una assurda violenza, alle torture alle quali è sottoposta una donna il cui unico reato è quello di avere combattuto per le sue idee, per una Bielorussia libera e democratica, e di non essersi mai piegata alla brutalità del dittatore. Consegno tale richiesta a lei, signor quella voce, resa inudibile dalla volontà del regime, trovi qui, in quest'Aula parlamentare, spazio, corpo, forza, resistenza, vita. *(Applausi)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere, per il suo tramite, con urgenza che il Governo, un Ministro o lo stesso presidente Meloni, venga a riferire in quest'Aula sulle troppe incertezze e le troppe voci che circolano sull'attuazione del PNRR. Dal PNRR dipende il futuro di questa Nazione, il futuro economico e sociale. Lo dite anche voi e l'avete scritto nel DEF: il 90 per cento del PIL dell'Italia nel 2024 dipende dal PNRR. Invece, non abbiamo nessun dato. Gli ultimi dati che abbiamo li abbiamo avuti tutti dal ministro Fitto o, ancora lo scorso *weekend*, dal *report* presentato dal Forum Ambrosetti. I dati non sono per niente per niente soddisfacenti, ma anzi sono allarmanti. Non solo si evince un ritardo cronico, ma anche che stiamo procedendo - così come detto anche dal *report* di Ambrosetti - a macchia di leopardo, direi anche a caso, tagliando di qua, spostando di là, con il risultato che molti progetti sono stati cancellati o - come direbbe il ministro Fitto - rimodulati, altri sono stati rimandati ad altra data da destinare, altri ancora hanno visto ridurre dimensioni e risorse.

dei progetti e, di quelli relativi all'inclusione e alla coesione, solo l'8 per cento. È questa l'eredità che ci sta lasciando il ministro Fitto alla vigilia della sua partenza per Bruxelles: un Ministro che ha cancellato l'Agenzia della coesione, che ha avocato a sé tutte tutte le deleghe e le competenze per il PNRR, per il Fondo sviluppo e coesione, per i fondi strutturali, per le ZES, e che cosa succede? Che fine faranno queste deleghe? Chi se ne occuperà? Questa è la mia richiesta per il suo tramite, perché altrimenti si rischia di non avere certezze, di non avere risposte e le incertezze sono tante. Ci siamo lasciati, alla chiusura dei lavori, con un ministro Giorgetti che chiedeva addirittura una proroga a Bruxelles; un ministro Fitto che in audizione ha anche detto che occorreva revisionare il PNRR. Il ministro Musumeci, in una intervista, dice che addirittura o si deroga al 40 per cento delle risorse destinate al Sud per i progetti dalla Protezione civile o viene rimodulato tutto il Piano a livello nazionale. Presidente, è davvero troppo, bisogna che questa Assemblea venga informata il possibile. E nel frattempo cosa succede in Europa? Ve ne siete accorti? Ursula von der Leyen ha dovuto rimandare la nomina degli ultimi elementi della Commissione, perché il ministro Fitto non convince, e almeno su questo eravamo d'accordo, perché non convinceva potrei continuare. *(Applausi)*. Questa Assemblea e il Paese chiedono risposte; ce le chiedono soprattutto i Comuni, che sono per la quasi totalità i destinatari dei progetti di attuazione, hanno aperto cantieri, hanno messo in campo professionisti e non hanno risposte. Anche in quest'ottica abbiamo abbiamo presentato il disegno di legge che prevede l'istituzione di una Commissione di vigilanza e il controllo sull'attuazione del PNRR. È una risposta che deve essere data non solo a quest'Assemblea, ma a tutto il Paese: è un piano che dovrebbe traghettare l'Italia a un futuro migliore,

«Onorevole Presidente, La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dal dott. Gennaro SANGIULIANO dalla carica di Ministro della cultura. Con il medesimo decreto il Presidente della Repubblica ha nominato il sig. Alessandro GIULI Ministro della cultura.